Signor Presidente, in data 30 marzo 2009, l'Assessorato alla sanità della Regione Umbria ha comunicato all'ufficio competente del Ministero, quale punto di contatto nazionale del sistema di allerta comunitario, l'avvenuto riscontro di particelle di natura metallica nel prodotto alimentare «Pappa pronta Mio verdure pollo e semolino» (lotto L 72500741) della Nestlè, nelle confezioni in vasetti di vetro da 250 grammi. Il prodotto risultava fabbricato in Germania e distribuito in Italia dalla Nestlè italiana Spa-Milano. La Regione ha comunicato, inoltre, che il campione è stato consegnato alla competente ASL dal nucleo mobile della Guardia di finanza Compagnia di Foligno. Relativamente alle misure adottate dalla ditta citata, l'Assessorato alla sanità della Regione Lombardia ha segnalato a questo Ministero che la ditta, oltre a fornire le liste di distribuzione, ha subito attivato le procedure per il ritiro del prodotto oggetto di allerta, pubblicando il *recall* anche su quotidiani a diffusione nazionale, quindi garantendo la più ampia informazione dell'avvenuto ritiro. Signor Presidente, vorrei ringraziare il sottosegretario Martini che ha inteso venire a rispondere in Aula, questa mattina, con una procedura estremamente veloce.

Lo dico anche perché il Ministero dell'agricoltura fa un'ampia diffusione di notizie relative alla tutela di questi prodotti.

non solo perché tocca da vicino la salute dei consumatori, ma anche perché oggi è un tema particolarmente sensibile nel consumo di determinati prodotti.

prodotto: non possiamo infatti parlare di filiera corta, né di prodotto biologico, né di garanzie di coltivazione quando apprendiamo che il prodotto è fabbricato altrove.

Signor Presidente, attualmente la rete italiana di banche di sangue cordonale è costituita da 17 banche distribuite su tutto il territorio nazionale. La rete di donazione, raccolta e *banking*, che ricomprende i punti nascita, le strutture trasfusionali e le unità operative di ematologia dove risiedono le banche, le unità di trapianto emopoietico e le Autorità competenti (Regioni, Centro nazionale sangue e Centro nazionale trapianti), si distingue per l'applicazione rigorosa dei requisiti di qualità e sicurezza introdotti dalla normativa italiana ed europea e per la partecipazione attiva ai *network* internazionali, con la specifica finalità di garantire un elevato grado di qualità e sicurezza delle unità cordonali destinate al trapianto emopoietico. L'elemento determinante per garantire la sicurezza del sangue cordonale è l'applicazione di rigorose procedure di selezione delle madri e delle coppie prima della donazione. Ciò comporta raccogliere un'attenta anamnesi fisiologica e patologica, sia familiare che personale della madre e del padre, ed escludere, in conseguenza di motivazioni cliniche documentate, tutte quelle donazioni che possano essere a rischio di trasmissione di patologie nel potenziale ricevente. La raccolta e la conservazione dedicate di sangue cordonale (nei casi previsti dall'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza ministeriale del 26 febbraio 2009) sono finalizzate al trattamento terapeutico di familiari, generalmente un fratello o una sorella che al momento della nascita risultano essere affetti da patologie, per lo più di carattere ematologico, per le quali è scientificamente dimostrata la necessità e l'appropriatezza dell'uso di cellule staminali emopoietiche nell'ambito di un trattamento trapiantologico. La conservazione dedicata, come prevista dalla stessa ordinanza all'articolo 1, comma 4, e come ricordata nel *dossier* «Uso appropriato delle cellule staminali del cordone ombelicale» citato nell'atto parlamentare, viene effettuata anche nel caso di famiglie ad alto rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate, per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale. In merito ai quesiti posti, preciso quanto segue. 3.167 unità sono state qualificate come idonee alla conservazione, in quanto rispondenti ai requisiti necessari per essere efficacemente utilizzate a scopo di trapianto emopoietico. E' da rilevare che l'indice di *banking* rispetto all'indice di raccolta è stato del 27,5 per cento, quindi superiore all'anno 2007, in cui tale indice era pari al 24,2 Il mancato bancaggio di circa due terzi delle unità è fisiologicamente conseguente alla necessità di garantire standard qualitativi e di sicurezza conformi alle norme nazionali ed internazionali. Peraltro, la percentuale italiana di mancato bancaggio delle unità non rispondenti alle specifiche richieste è sostanzialmente sovrapponibile a quella rilevabile in ambito europeo. Sono a disposizione degli onorevoli senatori i dati relativi alle unità bancate presso ogni singola banca nel 2008, in allegato alla risposta. la accettazione delle richieste di donazione. Nessuna unità donata raccolta in sala parto è rifiutata dalle banche pubbliche, in quanto non esistono motivi di rifiuto di una unità cordonale, una volta che questa sia stata raccolta e trasportata presso la banca. Tutte le unità cordonali che pervengono alle banche vengono sottoposte a controlli per valutarne le caratteristiche quantitative e qualitative. Se le unità non corrispondono ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dalla normativa vigente e dagli standard nazionali e internazionali, e di conseguenza non sono utilizzabili ad uso terapeutico, più frequentemente sono utilizzate per studi di ricerca o per la messa a punto di nuove metodiche e procedure. Nell'ambito del consenso informato la madre o la coppia sottoscrivono la propria autorizzazione a tale impiego, qualora l'unità cordonale non risultasse idonea al bancaggio. Il terzo punto riguarda le richieste di conservazione per uso dedicato.

il rilascio dei nulla osta decorre dal 2005, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale 7 aprile 2005, che prevedeva tale procedura; il numero di nulla osta rilasciati in tale anno, da giugno a dicembre, è stato pari a 28;

il potenziamento della rete di biobanche. In via preliminare, in merito al riferimento fatto dall'atto ispettivo in esame alle dichiarazioni del sottosegretario di Stato, onorevole Eugenia Maria Roccella, mi corre l'obbligo di precisare:

Piano sanitario nazionale, l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009 ha individuato l'utilizzo di una quota pari a 10 milioni di euro. Gli obiettivi di tale finanziamento dovevano essere definiti in progetti specifici da presentare entro il 25 maggio scorso da parte delle Regioni. Gli obiettivi specifici di tali progetti, in linea con i fabbisogni assistenziali nazionali ed internazionali, sono: aumentare sul territorio nazionale il numero dei punti nascita dove è possibile effettuare la raccolta; realizzare programmi di formazione e qualificazione del personale addetto

Tutto questo al fine di incrementare complessivamente l'inventario nazionale delle unità cordonali e di ampliarlo con un numero crescente di unità provenienti anche da minoranze etniche, stabilmente presenti nel nostro territorio, al fine di tendere ad un ottimale allineamento rispetto alle richieste terapeutiche. terapeutiche. Esiste, inoltre, un sostanziale consenso con le Regioni, finalizzato a razionalizzare le risorse mediante la creazione di reti integrate di raccolta sia a livello regionale sia interregionale, e che ha come obiettivo il potenziamento delle banche già attive. Non è peraltro prevista la creazione di nuove, con l'eccezione della Regione Sardegna; in questo caso infatti le autorità regionali hanno già dato l'autorizzazione in tal senso da considerarsi strategica in considerazione della situazione territoriale e della particolarità genotipica di tale popolazione.

lo sono state altrettanto, soprattutto nella parte in cui richiedevo dei numeri e i numeri sono stati forniti.

come si intende operare, da una parte per rendere più funzionali queste banche pubbliche - tra le quali è inutile citare i casi di Matera e Sciacca

di donazione e il numero effettivo di campioni conservati - lo sta a dimostrare: non importa per un sistema pubblico quanti sono i campioni, ma la qualità dei campioni che poi possono essere utilizzati per i trapianti. L'interrogazione presentata serviva proprio per fare

promuovono la donazione pubblica, come deve fare sempre di più l'Italia, però permettono anche la conservazione autologa e che il privato, in qualche modo, possa